L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

***Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

Signor Presidente, vengo a parlare oggi di un tema che è particolarmente rilevante sotto il profilo della tutela dei diritti umani e sotto il profilo del contrasto alla criminalità organizzata.

prima firma della senatrice Amati, un altro a firma della senatrice Carloni ed un altro, presentato da me, che riassume un po' il lavoro di cui mi ero fatta portatrice nella mia precedente esperienza esperienza come presidente della commissione interministeriale contro la tratta di esseri umani e capo dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Naturalmente, nell'ambito del mio disegno di legge cercavo di far convergere anche esperienze derivanti dalla mia attività di magistrato, che si era concentrata soprattutto sul contrasto alla criminalità organizzata e, per molti versi, al traffico degli esseri umani. esseri umani. Il ritardo con cui questa Convenzione viene ratificata lascia veramente perplessi, tenendo conto che la Convenzione di Varsavia recepisce sostanzialmente scelte normative e quindi dovrebbe essere motivo di grande soddisfazione per l'Italia che la propria legislazione venga presa in considerazione e a base di un provvedimento del Consiglio d'Europa.

tra i Paesi europei e consente di tutelare in maniera uniforme le vittime della tratta e, al contempo, di contrastare in maniera uniforme il fenomeno della tratta degli esseri umani sotto il profilo della penalizzazione dei trafficanti.

Nell'era del globalizzazione, caratterizzata da fenomeni ed esigenze complesse, che vanno dalla tutela dei diritti fondamentali dei migranti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico dei Paesi di destinazione, si viene a collocare una moderna forma di schiavitù, che riproduce a distanza di millenni l'equazione aristotelica tra asservito e barbaro e che è strumento di profitto di pericolose organizzazioni criminali transnazionali. umani costituisce una grave violazione dei diritti umani che si traduce nella mercificazione della persona, nella sopraffazione della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. Per tale ragione, le azioni di contrasto al fenomeno della tratta, quale che sia lo scopo di sfruttamento prefissato dai trafficanti (sessuale, lavorativo, espianto di organi), non possono che essere fondamentalmente orientate alla tutela dei diritti umani delle vittime; il momento dell'identificazione, assistenza e protezione sociale delle stesse costituisce l'asse portante di qualsiasi azione integrata di contrasto al fenomeno nella duplice ottica della repressione nei confronti dei trafficanti e del supporto e protezione sociale delle persone sfruttate. Questa ottica è al centro delle principali norme di carattere internazionale che i colleghi del Partito Democratico hanno già richiamato nei loro interventi e, per quanto concerne il nostro ordinamento giuridico, dello strumento costituito dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalle norme contenute nella legge 11 agosto 2003, n. 228, che recepisce la Convenzione di Palermo e i Protocolli allegati, prevedendo reati contro la riduzione in schiavitù e la tratta di persone. Il traffico di esseri umani come forma di grave sfruttamento coinvolge non solo adulti, soprattutto donne, ma anche minori, sia di genere femminile (in maggioranza) che di genere maschile, e una componente significativa di transessuali. Si tratta di un fenomeno plurale, soggetto a trasformazioni repentine sotto la pressione che le forze di polizia esercitano su di esso delle azioni di protezione sociale e di accoglienza che i servizi territoriali attivano in favore delle vittime; un fenomeno che si estende, interessando segmenti di gruppi nazionali diversi, con modalità diverse di coinvolgimento nella tratta e nello sfruttamento, ora manifeste, ora difficilmente individuabili, ora non espresse e mimetizzate proprio al fine di non essere comprese e contrastate. In generale, si tratta di un fenomeno transnazionale, gestito da organizzazioni senza scrupoli che operano tra i Paesi d'origine, quelli di transito e quelli di destinazione, e che oggi raggiunge profitti sempre più rilevanti. In effetti, come denunzia fortemente anche la Procura nazionale antimafia, la criminalità organizzata, attraverso lo sfruttamento del bisogno di opportunità di reddito, di lavoro, di una vita migliore di una popolazione vulnerabile, costruito, accanto al traffico di droga e di armi, un fiorente traffico di migranti, con ramificazioni e profitti sempre più estesi. Si calcola che i profitti siano inferiori soltanto a quelli del traffico di armi e di stupefacenti. Il Procuratore nazionale antimafia ha denunziato che la tratta rappresenta un fenomeno sempre in maggiore crescita, principalmente a causa delle condizioni di estrema povertà, al limite della sopravvivenza, in cui sono costretti a vivere gli abitanti di alcuni Paesi, del loro sfruttamento da parte di trafficanti senza scrupoli, che realizzano, in violazione dei più elementari diritti dell'uomo, una moderna forma di schiavitù con enormi profitti ed un alto tasso di impunità. Il traffico è ormai organizzato come una vera e propria impresa criminale, nella quale sono coinvolti tutti i livelli della criminalità, dai piccoli gruppi alle grandi reti internazionali degli stupefacenti e delle armi, e dove tutti si arricchiscono operando su diversi versanti con una ripartizione di compiti.

che dovrebbero richiedere un'attenzione precipua di tutto il Parlamento; invece, abbiamo attenzione se le leggi sono *ad personam*, se si instaura un dibattito a livello politico,

se non vogliono rimanere, come giustamente dice il Presidente, quanto meno di non distogliere l'attenzione di chi dovrebbe essere obbligato a sentire, non fosse altro che per la funzione di parlamentare e per l'impegno che dovremmo mettere in certi argomenti.

la prima ad evidenziare che per combattere le organizzazioni criminali vanno poste in essere contemporaneamente due azioni: non solo quella di perseguire i trafficanti, ma anche quella della prevenzione, tutela e assistenza delle vittime. Ciascuna azione se adottata da sola - dice il Procuratore nazionale antimafia - non è sufficiente. La repressione giudiziaria, se inefficace, si ripercuote negativamente anche sulla fiducia e sull'incolumità della vittima, che può addirittura subire vendette e ritorsioni dagli sfruttatori indicati e non perseguiti. D'altra parte, però, la mancata individuazione di persone come vittima di tratta e l'assenza di qualsiasi informazione impedirebbero alla radice la repressione dei reati che resterebbero, come spesso avviene, una realtà sommersa. Credo che sia una denunzia molto seria, anche perché proviene da una fonte molto qualificata. In conseguenza, nell'attuale momento storico non si può prescindere da un approccio al fenomeno della tratta degli esseri umani diverso da quello europeo e internazionale, ossia come espressione di una politica rivolta al contrasto della criminalità e al contempo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Questa strategia è espressa in maniera emblematica dalla Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e firmata dall'Italia l'8 giugno 2005, senza ancora che sia intervenuta la ratifica. La Convenzione, che - come dicevo - recepisce larga parte della legislazione italiana, denunzia il disvalore proprio del delitto di tratta quale grave violazione dei diritti fondamentali, ed in particolare della dignità, libertà ed incolumità psicofisica della vittima, e tende a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando al contempo i diritti delle vittime - in particolare quelli violati dallo sfruttamento sessuale - secondo un approccio non discriminatorio, attento sia alla prospettiva di genere (che spesso

In tale contesto si inquadra un efficace sistema di assistenza alle vittime del *trafficking*, che comprende la concessione *de iure* di permessi di soggiorno per ragioni umanitarie (come già previsto dall'ordinamento italiano di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al fondo per le vittime della tratta, già istituito, peraltro, dall'Italia con la legge 11 agosto 2003, n. 228. La Convenzione sancisce inoltre, in capo agli Stati firmatari, un obbligo di incriminazione Vorrei brevissimamente accennare, se il Presidente mi concede altri due minuti, qual è il nostro sistema e perché è importante che la Convenzione venga a completarlo. La La legislazione italiana si occupa di entrambi gli aspetti che ho richiamato, che riguardano il contrasto e la tutela delle vittime. Sin dalla sua entrata in vigore la legge italiana sulla tratta (parliamo del 2003), in piena sintonia con la Convenzione di Palermo e con il Protocollo annesso, anticipando anche i principi ispiratori della Convenzione del Consiglio d'Europa, ha utilizzato sia a livello penale che processuale tutti gli strumenti e le misure di contrasto già sperimentati la possibilità di concedere uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale allo straniero. A questo riguardo, il ministro Amato emanò una circolare molto importante, richiamando l'attenzione dei questori delle Province affinché ci fosse una distribuzione unitaria di permessi sul territorio nazionale e affinché questi permessi fossero effettivamente rilasciati. Purtroppo la circolare del ministro Amato, che fa riferimento anche a precedenti circolari di altri Ministri e a interventi del Capo della Polizia, non ha ricevuto un'adeguata applicazione,

Vorrei far presente che, secondo le stime prodotte dal Procuratore nazionale antimafia, i permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari e di protezione sociale ammontano, dal 1998 al 31 luglio 2008, a 3.919. Sono questi permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale che consentono alle vittime di tratta di diventare efficaci testimoni nei processi che si svolgono a carico dei trafficanti. Questo spiega perché il percorso sociale costituisce un ottimo strumento per poter sconfiggere la criminalità organizzata. Vorrei spiegare brevemente per quali motivi abbiamo inteso presentare emendamenti, alcuni dei quali riguardano una forma più efficace di contrasto al traffico di esseri umani e altri una tutela più adeguata delle vittime. Abbiamo previsto emendamenti che sono stati già in parte accolti dalla Commissione e abbiamo ritirato quelli che sono stati invece recepiti dalla recente legislazione, su proposta del Partito Democratico. Particolarmente importante sarebbe stata e sarebbe la presenza del Ministro per le pari opportunità in questa sede per la parte che riguarda la tutela delle vittime. Mi riferisco anche e soprattutto all'aumento dei fondi, che sono particolarmente ristretti rispetto al numero delle vittime ammesse ai programmi di protezione sociale, e quindi all'incremento delle risorse destinate al fondo per le misure antitratta e ai programmi di assistenza. Particolarmente importante sarebbe altresì il rilascio del permesso di soggiorno anche per favorire il ricongiungimento familiare. Al riguardo richiamo la

Naturalmente tutte le modifiche che proponiamo sono strettamente riconducibili alla stessa Convenzione di Varsavia, che prevede l'implementazione delle misure sia di contrasto, sia di tutela delle vittime.

L'argomento è balzato all'attenzione dei Paesi europei dopo il 1990, quando la caduta dei regimi comunisti

insieme a normali procedure, ha previsto recentemente un numero verde contro la tratta (e di questo va dato atto al Ministero delle pari opportunità)

che dovrebbe essersi avviato a partire dall'anno scorso. Sarebbe davvero interessante sapere quante scuole hanno messo in pratica quel programma e in quante scuole si sta veramente parlando di Costituzione e di principi. Questo sarebbe un dato interessante.

ha un sistema di protezione e di possibilità di protezione delle donne oggetto di tratta molto valido e all'avanguardia, che molti Paesi

in Macedonia, terra di transito della tratta delle donne moldave verso i nostri Paesi;

finanzia con fondi cospicui progetti di reinserimento delle vittime della tratta nei loro Paesi di origine. Personalmente, ho incontrato ragazze nigeriane che avevano scelto di rientrare nel loro Paese di origine e che, grazie all'Organizzazione internazionale migranti ma anche ad altre ONG

che molte ragazze manifestano la volontà di uscire da questo tunnel in cui sono finite, è anche vero

Siamo assolutamente convinti che sia necessario ratificare la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa: fortunatamente, il nostro Paese è, a mio avviso, tra i meglio attrezzati per recepirla

finalmente oggi si discute un atto particolarmente importante: un disegno di legge al quale sono anche molto legata, perché è stato uno dei primi che ho presentato in questa legislatura, come le mie colleghe Carloni e Della Monica, raccogliendo un testimone lasciato da altre nelle legislature passate. di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia quasi cinque anni fa; forse troppi, per un tema così significativo e, in teoria, di scontata condivisione tra le diverse forze politiche in campo. Nell'ambito delle convenzioni internazionali, se ci riferiamo al tema della schiavitù si può partire dal lontano gennaio 1815, dal Trattato stipulato nell'ambito del Congresso di Vienna e limitato alla tratta degli schiavi dell'Africa nera,

Seguirono le Convenzioni di Ginevra del 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e del 1933 per la repressione della tratta delle donne

Da qui verranno poi una serie di atti importanti, tra cui voglio ricordarne alcuni: il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1966 e ratificato nel 1977; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre del 1989 e ratificata nel maggio 1991; la Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 e ratificata nel 1998; la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, approvata nel dicembre del 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e adottata dalla stessa Assemblea generale nel febbraio 1995, sul traffico di donne e di ragazze. In questo percorso di atti ufficiali, volti nel tempo a riconoscere i diritti dell'uomo, della donna e del fanciullo, si legge la trasformazione negli anni del concetto stesso di schiavitù, così come del concetto di tratta, che ha acquisito una sua sostanziale autonomia; ne parlava bene ieri il senatore Di Giovan Paolo. La tratta oggi si può definire come il risultato di diversi eventi criminosi interconnessi: lo spostamento di una persona da un luogo diverso da quello di origine attraverso l'inganno o l'uso della forza per sfruttarne in diversi modi il corpo intero o parti di esso. Con l'espressione «tratta degli esseri umani», secondo la Convenzione che oggi dovremmo ratificare si designa «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o altre forme di coercizione, mediante rapimento, frode, inganno, abuso di autorità o situazione di vulnerabilità o mediante l'offerta o accettazione di pagamenti e vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento». Lo sfruttamento comprende, quanto meno, lo sfruttamento dell'altrui prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate - la questione del lavoro è un tema che spesso viene sottovalutato quando si parla di tratta -, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi. È evidente come è definito nell'articolo 4 della Convenzione, il consenso di una vittima allo sfruttamento prospettato è irrilevante quando sia stato usato uno qualsiasi dei mezzi coercitivi sopra enunciati. La vittima è la persona fisica sottoposta alla tratta e quando essa ha meno di 18 anni si parla di tratta di minori. Il fenomeno della tratta ha subìto una profonda trasformazione soprattutto negli ultimi decenni, quando la globalizzazione economica, lo sviluppo dei mezzi di informazione, la caduta del muro di Berlino, hanno favorito il movimento di centinaia di migliaia di persone. In queste condizioni, In queste condizioni, canali illegali, gestiti da gruppi criminali, hanno potuto trarre grandi vantaggi sfruttando le speranze dei nuovi migranti. Da qui prevalentemente si è conosciuta la prostituzione coatta, della quale le organizzazioni criminali gestiscono il traffico, definiscono il reclutamento, il trasporto e l'assoggettamento paraschiavistico delle vittime anche minori. Le modalità di reclutamento sono diverse, dal raggiro al reclutamento forzoso, al vero e proprio ricatto su di sé o sui propri parenti. Ciò che resta immutato, e che accade una volta reclutate le persone da trafficare, è che queste saranno soggette ad imposizione e mercificazione di loro stesse. Per questo è indispensabile che in ogni Paese ci sia un controllo sempre più serrato, si incrementino le risorse e le persone destinate ai servizi di protezione, si arricchisca la loro formazione professionale in modo da poter meglio identificare e sostenere le vittime. È evidente, inoltre, che l'apertura dei confini ha vastamente facilitato l'estendersi di questo fenomeno, con la conseguente necessità politica di collaborazione tra Paesi diversi, se si vuole cooperare per contrastare il fenomeno criminale da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, e se si vuole anche dare risposta alle vittime, sperando di poter realizzare forme di integrazione lavorativa. Molto è stato fatto con il passato Governo e con il lavoro del del nostro Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricordo anche il progetto «Equal Tratta No!»; ricordo i materiali da questo prodotti insieme all'AICCRE, anche di buona utilità. Bisognerebbe, però, sapere quanto e come questi siano stati poi di fatto utilizzati. Certo, dopo cinque anni, si sarebbe potuta auspicare l'approvazione di un disegno di legge più complesso, nel quale tenere in adeguata considerazione come ha suggerito la senatrice Della Monica durante la discussione in Commissione ‑ anche l'evoluzione giurisprudenziale sulle materie riguardanti soprattutto le modifiche all'articolo 600 del codice penale. In ogni caso, oggi, con la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea, Paese non solo ottempera finalmente ad un obbligo politico di ordine internazionale, ma soprattutto definisce uno strumento che speriamo sia efficace e che comunque è ineliminabile per tutelare adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

approveremo questo strumento di ratifica sarà una giornata importante per il Parlamento italiano, e mi auguro che da parte del Governo e della maggioranza non ci siano tentativi di dilazione. Finalmente verrà ratificata la Convenzione firmata ormai nel lontano 2005 e si porranno le basi per un'azione giuridica condivisa per la lotta alla tratta degli esseri umani. La schiavitù esiste. La schiavitù esiste. Questa è la tragica realtà con la quale dobbiamo misurarci, e non serve l'emozione superficiale di fronte a qualche frammentaria notizia o a qualche singolo caso, emozione che lascia presto lo spazio ad una sostanziale indifferenza. Sono passati poco più di 60 anni, signor Presidente, dal dicembre 1948, quando l'Assemblea delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la quale all'articolo 4 proclama: «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma». Eppure, la schiavitù esiste ancora. Dobbiamo purtroppo farcene In un interessante saggio del nostro collega senatore professor Livi Bacci si esplicita come in 400 anni, dall'Africa all'America, furono trasportati quasi 10 milioni di schiavi. Oggi, nel civile mondo globalizzato, si calcola che esistano almeno 27 milioni di schiavi. Certo, non è più una schiavitù basata sul possesso giuridico assicurato da una legislazione contraria ai principi di civiltà, ma è una schiavitù altrettanto crudele. È la schiavitù del debito, che asservisce milioni di esseri umani, per debiti a volte modestissimi secondo i parametri occidentali, di qualche decina di dollari, ma che si trasferisce di padre in figlio in una catena senza fine. È la schiavitù in qualche modo contrattualizzata, che noi abbiamo conosciuto a Rosarno, che nasce da un contratto di lavoro fittizio o da una promessa di un lavoro regolare in cui il nuovo schiavo viene di fatto sequestrato sequestrato e privato della sua libertà, con la minaccia di denuncia alle pubbliche autorità - perché quasi sempre è un immigrato clandestino - ed usato per lavoro nero o per prestazioni sessuali. Esiste perciò la schiavitù e, poiché siamo in un mondo globalizzato, lo sfruttamento della schiavitù migra dalle zone di reclutamento all'intero pianeta. La tratta degli esseri umani genera profitti paragonabili a quelli derivanti dal narcotraffico e dal commercio illegale di armi, con gravi conseguenze per la legalità e la sicurezza degli Stati, con una crescente capacità per i gruppi criminali di investire in ulteriori attività illecite o anche acquisire il controllo, con proventi illeciti, di istituzioni economiche e finanziarie. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono circa un milione gli esseri umani oggetti di traffico ogni anno nel mondo, e l'Organizzazione internazionale del lavoro stima in oltre 12 milioni gli individui sottoposti a sfruttamento lavorativo e sessuale: 12 milioni di cittadini di questo mondo. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne o ragazze, in più del 50 per cento dei casi si tratta di minorenni. Prostituzione, accattonaggio, lavoro nero costituiscono il mercato di sbocco per persone ridotte in stato di schiavitù e private di ogni diritto. Gli aspetti positivi della globalizzazione sono evidenti, con opportunità di crescita per aree finora escluse dall'accesso a beni fondamentali come l'alimentazione, la salute e l'istruzione. Tuttavia, è ancora inadeguata un'iniziativa multilaterale per combattere i due gravi squilibri che l'accompagnano: in primo luogo, l'accrescersi di profonde disparità di reddito all'interno dei Paesi e il permanere di sacche di povertà ed emarginazione assoluta (oltre un miliardo di esseri umani soffre la fame, ed il numero è in crescita); in secondo luogo, l'accrescersi della capacità di reti criminali transnazionali, che reclutano in fasce di popolazione senza speranza, a seconda del *business*, schiavi, spacciatori, lavoratori clandestini, manodopera per il terrorismo, e sono in grado di controllare il territorio di interi Stati e di costruirvi basi in grado di competere con le pubbliche autorità impotenti nella prevenzione e repressione. un'azione determinata a livello planetario, sia sotto il profilo della tutela dei diritti umani fondamentali, sia sotto il profilo della sicurezza globale. Vi è una evidente asimmetria tra il diffondersi di reti criminali globali e la capacità di un'adeguata risposta transazionale da parte degli Stati e delle organizzazioni sovranazionali. Per questo è importante la ratifica della Convenzione e mi auguro veramente che riusciremo a concludere questo processo in temi brevissimi. La legislazione italiana è in materia certamente avanzata, tuttavia è un segno di sottovalutazione e di distacco dalla comunità internazionale la mancata ratifica. La nostra ratifica servirà anche a sollecitare gli altri dieci Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata.

È necessario poi che tutti gli organismi previsti dalla Convenzione siano in grado di operare con autorevolezza e adeguata dotazione di mezzi, in considerazione del fatto che il fenomeno della tratta non solo si amplia, ma muta rapidamente luoghi, mezzi, organizzazioni. È anche indispensabile una adeguata azione di *intelligence* globale, e sottolineo in particolare la necessità di rendere pienamente operativo il gruppo di esperti GRETA, la cui istituzione è stata prevista dalla Convenzione. Naturalmente, e concludo, signor Presidente, il quadro normativo è solo lo strumento per un'azione preventiva e repressiva. Deve essere sviluppato con più ampiezza, come hanno argomentato anche i colleghi che mi hanno preceduto, il sistema dei servizi territoriali a disposizione delle vittime, in collaborazione con le forze dell'ordine, con organizzazioni non governative e con la rete dei poteri locali. Occorre un costante monitoraggio delle inchieste scaturite dalle denunce per realizzare mappe aggiornate delle reti criminali. È essenziale poi la gestione efficace dei programmi per assicurare il rientro volontario delle vittime ed il reinserimento nel Paese di origine, qualora lo richiedano. Infine, occorre sviluppare una azione culturale dì fronte all'opinione pubblica, che tende a vedere come un fenomeno unico fenomeni diversi: quello dell'immigrazione clandestina con propri mezzi, quello del traffico di migranti e quello della tratta. Non distinguendo i diversi fenomeni crescono sentimenti di paura per fenomeni non conosciuti, per le difficoltà di una integrazione con culture diverse, per i circuiti malavitosi che sempre si accompagnano alle diverse forme di illegalità che prosperano attorno ai movimenti migratori. Abbiamo il dovere di lavorare politicamente e culturalmente perché vi sia una piena percezione della gravità di questo crimine che entra come un cancro nel tessuto della convivenza civile. Non possiamo avere gli occhi spenti di fronte ad una violazione così grave dei dei diritti della persona. Con la ratifica faremo un passo in avanti importante, e questo è un bene per tutta la famiglia umana. Dichiaro chiusa la discussione generale.

D'altro canto, dal punto di vista della storia del diritto e dell'attenzione giuridica, la tratta degli esseri umani umani conquista un proprio profilo di sensibilità ed attenzione distinto dallo schiavismo per lo meno dal principio degli anni Ottanta,

Il fenomeno si lega non soltanto dal punto di vista dell'osservazione italiana ma di quella europea, occidentale, alla dissoluzione dei

necessario distinguere il profilo della tratta degli esseri umani dai tradizionali profili dello schiavismo schiavismo le abbiamo certamente, almeno in territorio italiano, con la dissoluzione della ex Jugoslavia. Chi ha cultura cinematografica ricorderà il bellissimo film "Vesna va veloce" che negli anni Novanta per poco non vinse a Venezia: trattava la storia di una giovane ragazza, istruita, coltivata, concepita e pensata per la prostituzione, che arriva in questo desolato territorio di una Romagna postfelliniana e viene palleggiata tra varie bande già insediate di criminalità organizzata e di un genere di criminalità organizzata del tutto distinto, seppur contiguo, da quello di cui ci siamo occupati ieri pomeriggio nella prima parte dell'ordine del giorno dell'Aula. Allora, da questo punto di vista, l'attenzione della comunità internazionale viene recepita proprio dall'organizzazione, se volete, in qualche modo, regionale delle Nazioni Unite che è l'OSCE, quella la cui antenata (la CSCE) aveva collocato quel terzo cesto dei diritti umani ai quali tende a rifarsi questo tipo di tematica, ed era stata in qualche modo alle origini della successiva distribuzione successiva distribuzione altrove di quei drammi che il comunismo non era più capace di nell'ambito del vecchio impero governato della vecchia Unione Sovietica. Da questo punto di vista, la Convenzione di Varsavia è stata molto interessante, molto sobria, ha cercato di sollecitare il minimo possibile di modificazioni dell'ordinamento interno. Da questo punto di vista - mi pare lo abbia notato stamattina la senatrice Della Monica, anche in Commissione particolarmente presente su queste problematiche

una cattiva volontà, una cattiva coscienza, da parte del Governo nel dare attuazione al provvedimento. Francamente - come affermato nella relazione che abbiamo preparato insieme al collega Benedetti Valentini e consegnato in Aula - assolutamente non si può dire che sia così.

il sottosegretario Caliendo ci ha annunziato che anche il Governo stava per intervenire. Non per questo, ben attenti all'autonomia dei profili parlamentari, ci siamo fermati, Benedetti Valentini ed io avevamo già fatto una prima relazione. Poi è sopravvenuto il provvedimento di questo Governo, il quale è stato assunto a testo base e di riferimento. Sui contenuti e sul modo di procedere, debbo ringraziare il senatore Perduca, che con molte citazioni in dettaglio ha riparato alla sensibilità ai tempi dell'Aula in funzione della quale noi avevamo invece ritenuto di allegare agli atti la relazione, peraltro già stampata. Ora, quello che emerge emerge in tutti gli interventi - alcuni forse non sempre di buon senso, non sempre di buon gusto nel loro pregiudizio antigovernativo (mi riferisco a quelli del senatore Pedica e di altri) - è che non abbiamo, come relatori, da replicare ad opinioni

come quella mediazione che ritenevamo con successo di aver raggiunto nelle Commissioni riunite grazie ad un ottimo suggerimento dell'ottimo sottosegretario Caliendo non sia stata sufficiente. Può darsi che, essendoci problemi di fondi, il Senato debba attendere il dopo Pasqua, e quindi la relazione della Commissione bilancio, per potersi pronunciare. Resta però un'indicazione che la senatrice Boldi ci ha dato e che mi consente di ritornare a quel bel film «Vesna va veloce». Certamente c'è

guarda alla sovrapposizione di questi temi quasi esclusivamente sul fronte libico come stazione di partenza: è difficile ritenere ritenere che le cronache possano dargli torto. Per quanto riguarda il resto della sovrapposizione (inevitabile e, come ho detto, più che legittima da parte dei colleghi dell'opposizione) fra le maglie dell'immigrazione «clandestina» (tra virgolette per la sensibilità di molti colleghi) o del permesso di soggiorno (in questo caso senza virgolette) e il profilo autonomo di ratifica della Convenzione, dobbiamo essere un pochino più sfumati. Non ci si può servire del momento di ratifica previsto nella nostra Costituzione in sede parlamentare per procedere a riforme di struttura dell'ordinamento interno.

apprezzare tutti gli interventi che sono stati formulati, e un po' di più quelli che hanno guardato al tema della tratta degli esseri umani sotto i profili di novità giuridica. Da questo punto di vista, credo che quella staffetta di buone intenzioni tra la più politica OSCE e il più giuridico - talvolta giuridicistico - Consiglio d'Europa debba trovare nel Parlamento italiano una pronta e immediata rispondenza, consapevoli (come più volte ci avverte il presidente Dini) che in questa materia i Parlamento, tendono a essere abbastanza biblici. In questo caso, lo sono stati un po' di meno, e non mi sembra di evocare esclusivamente

Credo che si vada verso un appuntamento successivo alla ripresa dei lavori, e mi riservo in quella sede, ove fosse necessario, di aggiungere qualche cosa e, diversamente, di pronunciarmi

una comune cultura giuridica e sociale di condanna di un fenomeno che rappresenta un'inaccettabile violazione dei diritti umani.

erano stati presentati ed erano all'esame della Commissione quando è intervenuto un disegno di legge del Governo che ha posto negli stessi termini una necessità

Governo, registrare questa comune volontà del Parlamento è già un grande successo, perché significa iniziare ad avere la cultura per combattere un fenomeno che nella nostra legislazione era già stato individuato. ma che oggi con la ratifica della Convenzione e l'ulteriore modifica del codice penale che viene proposta, credo possa essere uno degli obiettivi fondamentali del nostro Paese. Questa ragione mi porta a raccomandare che vi possa essere, anche in sede di votazione degli emendamenti, una unanimità di consensi.

Ho saputo, subito dopo, che essa era deserta perché era annunciato il «non voto», e la causa del non voto era la mancata presentazione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul provvedimento. Faccio fatica a pensare che questa mancata presentazione sia dovuta all'impossibilità o all'incapacità del Governo di

sulla quale il Parlamento ed il Senato in particolare sono stati richiamati più volte: per tre volte, con tre iniziative legislative da parte dell'opposizione, nel silenzio assoluto della maggioranza, fino a quando non è poi arrivato è poi arrivato il disegno di legge del Governo. Ho ascoltato con molta attenzione la discussione di oggi ed ho registrato che da parte della maggioranza ha preso la parola soltanto la senatrice Boldi, del partito del Presidente del Consiglio non hanno preso la parola sul provvedimento e, viceversa, l'opposizione ha espresso in modo chiaro le proprie opinioni, tanto da farle richiamare continuamente persino dai relatori. Presidente, intanto voglio esprimere il mio rammarico puntuale per la mancata la mancata ratifica di una Convenzione che tratta, come è stato detto da tutti in modo molto chiaro, di uno dei reati più abietti e più schifosi del nostro tempo, per il quale avremmo dovuto avere una fretta indiavolata nella ratifica, rispetto alla quale siamo esposti a sanzioni, critiche e osservazioni da parte di tutti gli organismi internazionali che si occupano della vicenda. Il Governo non vicenda. Il Governo non può oggi cavarsela dicendo che non votiamo perché non c'è la relazione tecnica del Ministero dell'economia. Il Governo deve impegnarsi

In secondo luogo, ritorno su un tema su cui più volte ho richiamato la Presidenza del Senato, e quindi, nuovamente, tramite lei, presidente Chiti, mi rivolgo all'intero Consiglio di Presidenza del Senato ed al suo Presidente. Questo è un ennesimo atto di svilimento delle funzioni del Parlamento, ed in particolare del Senato. Spero che anche i senatori della maggioranza si rendano conto di che cosa sta diventando il Senato della Repubblica. di Assemblea sono come questa. Io temo, signor Presidente, che tra poco verrà in mente a qualcuno di proibire le visite

un Senato nel quale il Presidente del Consiglio non ha più preso la parola dal giorno in cui è venuto a parlare per chiedere la fiducia al suo Governo; un Senato - me lo lasci dire, ma credo di poterlo dire a nome di tutti i senatori, compresi quelli della maggioranza: certamente della maggior parte dei senatori del mio Gruppo - nel quale anche i servizi

Senato, frequentare i luoghi dove ci si vede, dove i senatori discutono tra loro, per notare la rilassatezza dei servizi del Senato. Ma cosa vuol dire tutto questo? Possiamo noi continuare a lasciare senza commenti o osservazioni che il nostro lavoro sostanziale sia praticamente ed esclusivamente quello della conversione dei decreti-legge? Le interrogazioni parlamentari sono diventate dei

Le mozioni sono ormai calendarizzate in maniera bilanciata - una mozione di qua deve corrispondere ad una mozione di là in modo che la discussione si concluda con un voto dal quale emerga che la maggioranza è sempre maggioranza. Ma come possiamo pensare che questo sia il Senato di una Repubblica parlamentare?

da dove queste cose si dovrebbero vedere meglio e da dove si hanno anche i poteri per poter rimediare a queste condizioni.

io, da parte nostra, almeno nei confronti del senatore Zanda, dobbiamo dichiararci non colpevoli per aver commesso il fatto, e non per non averlo commesso. Voglio dire cioè che i lavori nelle Commissioni riunite sono andati come sono andati: c'è stata tutt'altro che sciatteria e insensibilità da parte della maggioranza, del Governo e del rapporto tra il Governo e la maggioranza! Non entro nella contabilità di precedenti legislature sulla maggiore o minore attenzione alla odiosità e alla schifosità - consideriamolo lessico extraparlamentare - della tratta degli esseri umani; quando colleghi che hanno lavorato fianco a fianco con noi - la senatrice Della Monica *in primis* - ci annunciano anche in Commissione che, per quanto apprezzassero il nostro nostro emendamento di mediazione, suggerito dal Governo e fatto nostro (soprattutto dal senatore Benedetti Valentini, che in materia di aggravanti si muove molto meglio di me), ritenevano alcuni profili estranei alla ratifica, ma di approfondimento strutturale dell'adeguamento interno, talmente importanti

e anticipare quella richiesta di ritiro degli emendamenti che, semmai, e soltanto dopo avere acquisito quegli elementi in seno alla Commissione bilancio, può chiedere il Governo. Elementi, però - mi permetta il collega Zanda - che per quanto riguarda la ratifica, così come prevista dal nostro ordinamento costituzionale,

quali, quanti e come sono i capitoli di bilancio che coprono questo problema: protezione sociale nel Paese di partenza, che magari non è la Moldova, ma è la Macedonia, anche per le moldave, anche come la problematica del permesso di soggiorno e dell'immigrazione clandestina possa ritrovare ritrovare qui dei punti di connessione. Pertanto mi sembra del tutto improprio considerare una sciatteria dell'Esecutivo e del rapporto tra il Governo e il Parlamento non essersi

Ci sembrava che l'esigenza di rispettare i disegni di legge dell'opposizione, quindi di rispettare il calendario, anche in presenza di un testo del Governo assunto come testo base, dovesse prevalere sull'esigenza procedurale procedurale della relazione e sull'attesa per l'esame di merito in Commissione. Per quanto riguarda l'amico Benedetti Valentini e me, ci sarebbe sembrato a dir poco scortese, se non antiparlamentare, iniziare i lavori ieri pomeriggio con quella insistenza al ritiro degli emendamenti che avrebbe consentito questa mattina di concludere. Peraltro credo che la Presidenza abbia valutato come l'appello del senatore Zanda al primo giorno utile non faccia perdere neanche ventiquattro ore alla delibera del Senato su questo provvedimento.

per rispondere appena in una battuta; lo faremo poi alla ripresa post‑pasquale, e lo faranno anche, credo, i membri del direttivo del mio Gruppo, con altra autorevolezza e competenza istituzionale. Approfittiamo della provocazione del sempre attento e incisivo capogruppo Zanda su questo argomento, che forse meriterebbe una discussione e un dibattito tematico. Lei, presidente Zanda, ha approfittato di questa occasione, come del resto è legittimo, per fare un affondo non lieve su un argomento straordinario, che è quello che riguarda la centralità del Parlamento, il suo ruolo, il suo rapporto con l'Esecutivo anche con altri mondi, con il dibattito politico in generale. Le posso dire, *apertis verbis*, a titolo personalissimo (poi, come ripeto, interverranno i nostri Capigruppo, che sanno quello che debbono risponderle),

vi ha risposto con grande puntualità e fondatezza il senatore Compagna. Io stavo semplicemente facendo il mio dovere, anche di garbo parlamentare, nel raccogliere la provocazione politica e istituzionale del senatore Zanda, per dare una prima, sommaria risposta: quindi, se lei crede che io sia fuori tema, debbo dirle che è fuori tema e intempestivo lei. Detto tutto questo, ben venga la provocazione. Se l'osservazione provenisse da un parlamentare di fresca nomina o da un politico

con qualche legislatura sulle spalle e qualche esperienza, qualche volta entusiasmante, qualche volta sofferta, a questo riguardo, debbo rispondere che questo scivolare del Parlamento fuori dal baricentro istituzionale e politico non risale certo all'altro ieri o all'inizio di questa legislatura. Penso che osservazioni di questo genere, ormai da diverse legislature, nel ruolo alternante di opposizione e di maggioranza, le abbiamo fatte in entrambe le Camere parlamentari. Ciò dimostra che questa è questa è una situazione che merita di essere affrontata, e se qualcuno pensa di andare per scorciatoie - lei sa a chi mi riferisco - attraverso bozze di riforma che prevedono direttamente la cancellazione del Senato come Camera parlamentare a sovranità popolare,

sia anche i lineamenti di rilievo costituzionale (che richiedono i tempi e gli approfondimenti propri di quella sede), sia un dibattito politico in senso stretto. Mi permetto di opinare,

anche il tipo di soglia e di livello di scontro politico, perché è di tutta evidenza che, negli schieramenti di maggioranza e di opposizione, si alza o si abbassa il livello, l'eclatanza, la durezza e la tenacia dello scontro a seconda di quanto anche l'opposizione voglia deliberare in ordine ai suoi comportamenti. Certo, se l'opposizione decide di utilizzare, come è legittimo, le sedi parlamentari allo stesso modo, né più né meno, di quelle non parlamentari, per una forte azione di denuncia, spinta fino all'ostruzionismo, è chiaro che la maggioranza e l'area governativa tendono ad adottare quei provvedimenti che garantiscano, comunque, l'attuazione del proprio programma. Invece, se si instaura un clima di natura diversa, allora vi sono altre strade, dettate più dalla politica

della maggioranza parlamentare con l'Esecutivo, che deve essere un rapporto proficuo, con l'opposizione ma, più vastamente, con l'opinione pubblica. Concludo ricordando che pochi giorni fa ho raccolto lo spunto di un altro provocatore intellettuale di prima autorità, il senatore Li Gotti, il quale parlava del modo giusto di legiferare e del modo cauto di produrre normative che fossero coerenti anche nella loro stesura.

forse un bene che tutti noi assumessimo uno stile meno congestionato, meno gridato, meno propagandistico, cercando di approfondire l'essenziale per arrivare a una legislazione di buona qualità, profondamente pensata prima di essere licenziata, perché questo non può che farci del bene. Notavo, inoltre, che da questo punto di vista anche il bicameralismo, quand'anche fosse tutto da migliorare,

sia al Senato che alla Camera, in virtù dei quali l'attuazione di principi costituzionali non determina la necessità della presentazione della relazione tecnica, perché l'attuazione della Costituzione deve trovare comunque, obbligatoriamente, la copertura in bilancio.

fossero specificatamente presentate, come richiesto dalla legge di contabilità, con il bollino della Ragioneria dello Stato. Trattandosi di una richiesta di tipo tecnico, non ha potuto che essere ricevuta dal Governo. Ma una relazione tecnica, che a questo punto non trova più precedenti per la rinnovata legge di contabilità, ha bisogno di qualche ora di tempo per essere predisposta. Quindi, le osservazioni del senatore Zanda sono in contraddizione con il fatto che è una giusta richiesta della minoranza che determina lo scivolamento di ventiquattro ore nell'approvazione del disegno di legge. Parlo di ventiquattro ore perché, trattandosi comunque

disposizione degli individui oggetto della Convenzione. Da ultimo, fare di ciò argomento per

Presidente, la trattazione di questo disegno di legge - mi sia consentita una piccola parentesi prima di avviarmi

tratta veramente del frutto di un lavoro organico, articolato ed armonico di tutte le forze che siedono in Parlamento.

assolutamente armonico per la realizzazione di un documento legislativo che interpreta le esigenze più avvertite dell'avvocatura italiana.

alla realizzazione di questo nostro prodotto attraverso una serie di audizioni - ce ne sono state più di una

affermare - credo di non fare torto a nessuno - che questo documento è frutto di una elaborazione allargata. stato sì costituito un Comitato ristretto, che ha lavorato in maniera agevole e snella - come avviene di solito quando i Comitati ristretti si costituiscono - ma è anche vero che l'interlocuzione con le aree più varie sotto il profilo culturale dell'avvocatura è stata sempre costante. Il documento che oggi ci apprestiamo a discutere, e a modificare nelle parti in cui lo riterremo necessario, è veramente il frutto di un impegno congiunto, di una elaborazione allargata, di una partecipazione avvertita. Ognuno dei protagonisti si è reso interprete delle esigenze dell'avvocatura e ha cercato di dare il proprio contributo. Posso affermare che il documento finale è di grande soddisfazione. È accaduto qualcosa, signor Presidente, che a mia memoria - ormai da qualche anno siedo in questi banchi - non ricordo sia mai avvenuto prima. Addirittura il Consiglio nazionale forense, l'organo istituzionale più alto dell'avvocatura, ha ritenuto doveroso e opportuno - questo ci lusinga molto prendere una intera pagina di grandi quotidiani a tiratura nazionale per dire che il documento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato riguardante il

Però, onorevoli colleghi, prima di addentrarmi, sia pur fugacemente, sugli argomenti portati dal documento che costituiscono questa grande innovazione, questa grande modernizzazione, fortemente voluta dall'avvocatura, debbo ricordare, perché lo reputo doveroso, un nostro collega che di questa iniziativa si è reso promotore in un momento difficile, nella scorsa legislatura, quando gli orientamenti più avvertiti ritenevano che si dovesse trattare della legge di riforma dell'avvocatura nel quadro

del senatore Guido Calvi, giurista illustre, che ha onorato per un lungo periodo il Senato della Repubblica, il quale, difendendo con grande vigore e grande capacità le prerogative che derivano all'avvocatura dall'articolo 24 della Costituzione (l'inviolabilità del diritto di difesa), sostenne, ed a ragione, che un tema che riguarda un ordine professionale professionale che si occupa di un diritto citato dalla Costituzione merita una trattazione assolutamente autonoma perché particolari e peculiari sono le esigenze che devono essere prese in considerazione,

questo riferimento a chi è stato il propulsore di tale iniziativa che adesso, nel corso di questa legislatura, ha trovato la sua considerazione più compiuta. Devo poi ringraziare in modo particolare tutti i membri del Comitato ristretto. Discussione equilibrata sempre, attenta sempre, propositiva sempre, quella che nell'ambito del Comitato è stata fatta: quindi, meritevole del rispetto e dell'ossequio da parte del relatore.

antica perché, da quando ci sono regole alle quali gli uomini si debbono uniformare per la convivenza civile, vi è sempre un avvocato che deve tutelare i principi tutelare i principi - che aveva bisogno di essere resa più adeguata e più coerente alle esigenze dei tempi, che si muovono freneticamente. La tutela dei principi è immutabile, è sempre la stessa: i principi non si toccano; però, le regole che accompagnano la tutela dei principi debbono essere naturalmente adeguate alle esigenze più avvertite. Già i criteri di accesso alla professione, onorevoli colleghi, sono stati rivisitati. Vedete, una realtà umana che supera ormai, sia pure di poco, le 200.000 unità si deve imporre dei criteri selettivi rigorosi: certamente, più rigorosi rispetto a quelli che finora hanno governato il sistema. È vero che la selezione nelle attività liberali dipende dalle capacità di chi le esercita e dal rapporto che si riesce a realizzare nei confronti della società, e che si costituiscono rapporti di apprezzamento che sono l'elemento più idoneo alla selezione, ma è altrettanto vero che bisogna verificare la sussistenza di taluni requisiti fondamentali. E allora il disegno di legge ha inteso riconsiderare i titoli di accesso, utilizzare strumenti più moderni e nello stesso tempo sottolineare come, fin dal primo approccio con l'attività professionale, si debba si debba dar prova di avere quelle attitudini e quella capacità per lo svolgimento dell'attività in futuro. Quindi, non più i vecchi compiti, come originariamente considerati, il vecchio tema sulle materie che venivano scelte, bensì

Il cittadino che va dall'avvocato deve avere la consapevolezza piena, al di là delle sintonie che si costituiscono sul piano umano, personale e culturale, che oggettivamente quel soggetto al quale affida i propri interessi, di qualsivoglia natura, si sottopone periodicamente a verifica della sua capacità.

ricorso a questo malvezzo abbiamo anche individuato dei criteri di ricognizione periodica che consentano di dire a coloro che l'avvocato non lo fanno, ma che egualmente

per la quale debba restare iscritto all'albo ed il regime delle incompatibilità che abbiamo disegnato contribuisce, a mio avviso in maniera sensibile, alla realizzazione di questa esigenza. Così come la tutela dell'assistito è garantita dall'assicurazione obbligatoria: gli avvocati dovranno adesso essere assicurati.

Un ultimo argomento, e poi mi avvio alla conclusione, sottolineando ancora una volta che all'esito della discussione generale sarà mia cura replicare a tutti i colleghi che riterranno di dovervi partecipare. Un Un argomento che mi auguro non appaia inelegante, perché è importante: quello della reintroduzione delle tariffe minime. Onorevoli colleghi, in ragione di normative forse troppo frettolosamente avviate si erano cancellati gli onorari minimi per gli avvocati creando una situazione disagevole di grande evidenza, ad una inelegante competizione al ribasso, realizzando una serie di proposte sempre meno qualificate dal punto di vista delle esigenze di natura economica, che inevitabilmente hanno comportato disagi per larga parte della nostra categoria. Ma quello che è più grave è che taluni soggetti, soprattutto le grandi realtà imprenditoriali e sociali, hanno hanno utilizzato nel loro esclusivo interesse questo stato di cose imponendo tariffe che certamente si si pongono su un piano conflittuale rispetto al decoro che un avvocato deve mantenere nel momento in cui in cui svolge la sua professione. L'avvocato deve avere consapevolezza del contributo che egli dà alle ragioni che gli vengono rassegnate e deve reclamare il giusto compenso; un giusto compenso che deve incontrare dei limiti nelle valutazioni che poi vengono fatte dal Ministero: perché le tariffe non le fanno gli avvocati, le tariffe le fa il Ministero. Questo aspetto pratico, che certamente non si può inserire nel novero de grandi temi che riguardano le vicende dell'avvocatura, è stato oggetto negli ultimi anni di grande fibrillazione all'interno dell'avvocatura stessa e di grande tensione; si sono dissolti una serie di rapporti con i grandi enti, si è creata veramente una situazione di grave disagio, di grave imbarazzo. Noi ci auguriamo che l'impianto che abbiamo ipotizzato possa intervenire e intervenga sulla materia e risolva questo problema; auspichiamo che venga riconosciuto all'avvocato almeno quel compenso minimo proporzionale all'impegno che egli dispiega. Onorevoli colleghi, mi fermo qui, ringraziandovi per la pazienza. Questa relazione, e l'avvio della trattazione di questo provvedimento, era attesa. L'avvocatura aveva anche avviato nei giorni scorsi qualche iniziativa di natura critica per le ragioni per le quali l'*iter* del disegno di legge non era stato ancora avviato. Adesso abbiamo cominciato e andremo avanti; l'auspicio è che l'*iter* si possa concludere entro il più breve tempo possibile. L'avvocatura italiana ha diritto a una normativa moderna e attuale, necessaria perché possa al meglio svolgere la propria attività.